vorrei ricordare come oggi il Parlamento sia chiamato a esaminare la relazione presentata in data 19 dicembre 2016 dal Governo alle Camere, relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con il fine proprio di aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Come è noto, la norma prevede, ai commi da 1 a 3, che, qualora il Governo, al fine di fronteggiare eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico di finanza pubblica, presenti alle Camere, una volta sentita la Commissione europea, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici e avanza una specifica richiesta di autorizzazione, che deve indicare la misura e la durata dello scostamento dagli obiettivi prefissati, oltre che definire il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Per eventi eccezionali, la stessa norma definisce periodi di grave recessione economica, come - ad esempio - recessioni che colpiscano l'area dell'euro o l'intera Unione europea o, allo stesso tempo, eventi straordinari che siano al di fuori del controllo dello Stato, come gravi crisi finanziarie che possono aver ripercussioni rilevanti sulla situazione finanziaria del Paese. Il comma 6 della stessa norma stabilisce che tale procedura si applica anche qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie, al fine di far fronte agli eventi eccezionali. È proprio questo il caso che esaminiamo oggi. La relazione presentata dal Governo fa specifico riferimento a questa circostanza, prefigurando un possibile intervento per un importo massimo fino a 20 miliardi di euro da reperire attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico. I presupposti di tale intervento vengono ravvisati nell'eventualità

stessi *test*, una carenza di capitale in presenza di scenari avversi; una carenza che - sottolinea la relazione - potrebbe risultare difficile da ripianare solo sul mercato sia per le presenti condizioni dei mercati finanziari, sia per la consistenza dei crediti deteriorati determinatisi in seguito alla recente e prolungata crisi economica e finanziaria. In altre parole - questo è importante sottolinearlo - pur nel riconoscimento che il sistema bancario italiano sia complessivamente solido e, quindi, non corra il rischio di crisi sistemiche, nella relazione viene riconosciuta la possibilità di alcuni casi ben individuati di crisi, che possono essere affrontati certamente con strumenti di mercato, ma allo stesso tempo possano prevedere un intervento pubblico. In altri termini, in alcuni di questi casi se il mercato non dovesse bastare, il Governo vuole garantirsi le risorse per poter varare una sorta di rete di sicurezza pubblica, onde evitare la risoluzione degli enti bancari ai costi drammatici che essa potrebbe comportare. Dobbiamo anche ricordare che il superamento delle crisi di alcune aziende di credito attraverso anche l'intervento pubblico potrebbe giovare non solo al complesso delle attività produttive del Paese, restituendo vigore alla funzione di intermediazione finanziaria del sistema bancario, sistema bancario, ma anche agli stessi risparmiatori, inclusi coloro che dovessero investire in azioni di banche avviate verso il risanamento e quindi in grado di realizzare nuovamente buoni profitti. In tutti questi casi di crisi, alla luce di quanto prevede la direttiva n. 59 del 2014 dell'Unione europea,

uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente bancario, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito negativo di prove di stress test che sono solitamente basati su scenari relativamente restrittivi e sono svolti dall'Autorità di vigilanza. Quindi, in seguito all'esito negativo di questi *stress test* e con la necessità di preservare la stabilità finanziaria, in un contesto quindi di possibile crisi sistemica, l'intervento pubblico vuole supplire alla deficienza dello stesso ente bancario e alla possibilità di raccogliere capitale sui mercati privati. Quindi, conformemente all'articolo 32 contenuto in quella direttiva, in questi casi si vuole evitare una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria attraverso la concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima e, quindi, in base alle condizioni previste da quella direttiva. La misura contenuta nella relazione si basa su due pilastri: il primo è una garanzia di liquidità per ripristinare la capacità di finanziamento a medio e lungo termine delle banche; il secondo prevede un programma di rafforzamento patrimoniale delle stesse banche nel rispetto delle regole dell'Unione europea. Il primo pilastro è relativo a delle garanzie su emissione di debito e rientra nella cornice normativa dell'Unione europea che mesi addietro ha autorizzato lo Stato italiano a fornire garanzie su liquidità sino a 150 miliardi di euro. Questo tipo di garanzia rappresenta per il debito pubblico una sorta di passività contingente - si potrebbe dire - suscettibile cioè di divenire tale. La seconda gamba, vale a dire il programma di rafforzamento patrimoniale, è relativa all'assunzione di partecipazioni dirette nelle banche dopo che è stata applicata la regola del *burden sharing*, e cioè il parziale sacrificio dei risparmiatori privati, a mezzo - ad esempio - di conversione in azioni del debito subordinato da essi detenuto. La relazione presentata dal Governo ribadisce la finalità precauzionale dell'intervento ipotizzato e precisa che esso non può essere al momento ancora dettagliato sia nei tempi, sia nelle modalità, sia nei singoli provvedimenti nei quali si articolerà. caso, risulta finalizzato ad assicurare due obiettivi di fondo: un adeguato livello di liquidità al sistema bancario e allo stesso tempo un rafforzamento patrimoniale delle banche medesime. Per il conseguimento di tale obiettivo, il Governo intende ricorrere a operazioni di emissione di titoli del debito pubblico fino ad un importo complessivo massimo di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 al fine di reperire le necessarie risorse. Si tratta naturalmente di un ammontare significativo di risorse, le quali tuttavia servono proprio a far capire a investitori e mercati che nessuna banca nel nostro Paese che presenti requisiti di solvibilità verrà avviata a risoluzione, in altre parole verrà lasciata fallire. È altresì evidente che potranno essere utilizzati molto meno dei 20 miliardi preventivati, anche perché quello che si potrà verificare e in parte si sta verificando - è che gli investitori, una volta compreso il quadro di interventi programmati, potrebbero trovare nuovamente conveniente investire ai prezzi correnti

confermato da un andamento relativamente positivo nelle ultime settimane dei titoli bancari quotati. Certo, va ribadito che è altrettanto importante, insieme al rafforzamento patrimoniale delle banche in crisi, in crisi, favorire ristrutturazioni, fusioni, razionalizzazioni, oltre che soluzioni dei problemi strutturali delle stesse banche. Molti di questi problemi in realtà sono non solo italiani, ma sono condivisi da altri sistemi bancari europei: si chiamano bassa redditività, eccessiva frammentazione, modelli di *business* in larga parte obsoleti, da rivedere e rilanciare. È quindi importante che, nel concedere l'autorizzazione, si riconosca che ricapitalizzare senza ristrutturare non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di un vero risanamento. Quindi, accanto alle operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario, finanziario, è necessario che vengano associati precisi impegni da parte delle banche nella riorganizzazione e ristrutturazione delle loro attività. Per tornare alla relazione, essa osserva che eventuali nuove emissioni di titoli del debito pubblico finirebbero per modificare sia gli obiettivi programmatici di fabbisogno e debito pubblico, approvati nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2016, sia il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato fissato nella legge di bilancio 2017;

nostro saldo e, quindi, di diminuzione dello *stock* di debito pubblico. Da ultimo Da ultimo è importante segnalare che l'ammontare degli effetti che in concreto si determineranno in conseguenza delle operazioni di emissione ipotizzate dal Governo, effetti sugli obiettivi programmatici sia di fabbisogno sia di *stock* di debito pubblico rispetto a quelli indicati nel DEF e nella legge di bilancio,

Sono in entrambi i casi delle grandezze da specificare una volta che si sarà delineato in concreto l'intervento da realizzare in favore delle banche in crisi. Per concludere, va ricordato come interventi di questo genere, vale a dire un intervento pubblico nel patrimonio di banche in crisi così come nel rifinanziamento di queste banche, che hanno interessato altri Paesi prima di noi (cito, ad esempio, i casi degli Stati Uniti e della Svezia), una volta che hanno determinato le condizioni di un rientro

all'indebitamento al fine di fronteggiare eventi straordinari è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Ricordo che i tempi del dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Dichiaro aperta la discussione.

consenso al provvedimento di autorizzazione alcune riflessioni che attengono all'esigenza, più volte richiamata, di una normativa organica in materia di credito e di gestione del sistema finanziario.

di riferimento che sia intelligibile non solo agli operatori finanziari e agli esperti della materia, ma anche e soprattutto ai cittadini

in funzione del compito che deve esercitare di sostegno all'economia e all'impresa. Diversamente, faremmo operazioni di salvataggio che rimangono ferme in una sorta di fotografia dell'esistente, che non attiva alcun tipo di rientro operativo sano del sistema a favore dell'economia, del rilancio dell'attività d'impresa e dell'occupazione. Penso, signor Presidente, che questo sia un tema che il Governo debba cominciare ad affrontare.

in una successiva legislatura. Noi, però, dobbiamo cominciare a rendere visibile, anche sotto il profilo normativo, qual è il funzionamento del sistema finanziario, del credito e delle banche, quali sono le garanzie a cui il cittadino può fare riferimento quando deposita i propri risparmi nella disponibilità di quel sistema, quali sono i servizi, i loro costi e come possono essere resi al massimo idonei al rilancio della nostra economia, che è già - come si sa - da tempo in una condizione di crisi.

nell'intervenire, perché mi sono stati riservati quattro minuti su un provvedimento di 20 miliardi di euro che è stato proposto in tutta fretta per risolvere una situazione, quella del sistema bancario italiano, giunta al limite del collasso.

con il Parlamento, affinché un atteggiamento di questo tipo non abbia più a ripetersi in futuro. Perdiamo ore e ore in discussioni inutili ma, quando si tratta di parlare di miliardi di euro, che sono il frutto del sudore di milioni di italiani, dedichiamo un tempo davvero infinitesimale.

da quello che ieri sera ha detto il cardinal Bagnasco in occasione della messa per le festività natalizie nella basilica di Santa Maria sopra Minerva:

stato oggi in discussione al Senato e ha voluto lanciare un richiamo a tutti noi. Il problema delle banche doveva essere affrontato alcuni mesi fa. Tutti i Gruppi politici avevano presentato la richiesta dell'istituzione di una commissione d'inchiesta per studiare la condizione del sistema bancario italiano. Invece abbiamo fatto fallire quattro banche anzi sei, se includiamo anche la Banca Popolare di Vicenza e la Banca Veneta - e oggi siamo qui a predisporre un provvedimento che riguarda una montagna di miliardi che non ci sono, perché la provvista doveva essere effettuata a debito, per risolvere una situazione che è arrivata al collasso. E mi crea anche un certo disappunto

però subito dopo che, senza un intervento precauzionale, il sistema creditizio potrebbe subire danni incalcolabili. Mi pare ci sia una contraddizione nel suo intervento.

costituzionale, per cui questo argomento scottante non ha potuto essere messo sul piatto. Siamo a 20 miliardi di ulteriore debito.

i diversi Governi - questo è il terzo - avvicendarsi a emanare provvedimenti a favore delle banche. Peccato che non siete mai stati in grado di risolvere il problema del sistema bancario italiano: anzi, lo avete peggiorato. La crisi del sistema bancario italiano non dipende solo dalla crisi economica che ha colpito Il problema della crisi bancaria italiana è la mala gestione delle banche italiane. E qua ci siete di mezzo voi, c'è di mezzo la politica, con gli interventi che ha fatto fuori dalla politica e con gli interventi fatti attraverso la politica. Avete fatto il decreto-legge IMU-Bankitalia cercando di ripulire i bilanci delle banche, ma non ci siete riusciti. Noi da circa quattro anni vi stiamo mettendo in guardia sul sistema bancario, ma voi siete andati avanti, avete continuato.

oggi voi venite qua a chiedere 20 miliardi per intervenire sul sistema bancario italiano, senza alcun piano. Non avete idea di cosa potete fare. Continuate a mettere toppe su toppe, come quella delle DTA,

darvi una cambiale in bianco, una carta di credito che potete spendere dove volete per 20 miliardi di A volte ci sorge il dubbio se siete incapaci o in malafede, perché noi che siamo gli siamo gli inesperti, quelli arrivati dalla strada che non sanno nulla di come funziona il mondo, vi avevamo messi sull'avviso vi avevamo chiesto di realizzare un piano perfetto per mantenere la fiducia degli italiani nel sistema bancario. Invece no! Il ministro Padoan,

Presidente del Consiglio invitava i cittadini ad investire nel Monte dei Paschi di Siena. Questo è il risultato: dobbiamo intervenire sul Monte dei Paschi di Siena. Ancora, in questa relazione non dite nulla anzi, se la si legge per bene si capisce che l'unico intervento pubblico che può fare lo Stato è quello che avviene dopo

che ora siete tanto spaventati da cosa potrà accadere al sistema bancario italiano. Il 4 dicembre avete ricevuto 20 milioni di no,

a dire che condivido la scelta che farà il nostro Gruppo, con grandissimo senso di responsabilità. Tuttavia il nostro voto, volto a portare avanti questa opera di razionalizzazione,

cito le responsabilità pregresse del Governo dimissionario in materia bancaria: nessuno dimentica i sospetti di *insider trading* che gravano sul dottor Carlo De Benedetti e su altri banchieri, che che - dicono le cronache - avrebbero avuto notizie anticipate sul famoso decreto-legge sulle banche popolari: procure della Repubblica, a che punto stanno le indagini su Carlo De Benedetti e su altri, visto che si parla di salvare le banche il cui fallimento sarebbe talmente disastroso che tutto il Parlamento è qui oggi riunito, in prossimità del

di quei risparmiatori che sono stati truffati facendo comprar loro titoli e anche modificando i loro profili bancari, trasformandoli in *rider* della finanza a loro insaputa. Vorremmo altrettanta rapidità per questi rimborsi. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi di Siena, cari colleghi, non non dimentichiamo la turpe storia targata PCI, PDS, PD e dintorni, i 28 miliardi di euro di sofferenze: soldi che sono stati dilapidati dalle gestioni politiche di sinistra del Monte dei Paschi di Siena. È una vergogna nella storia italiana che infama un istituto bancario che ha secoli di storia, che doveva essere un vanto dell'Italia e della storia economica dell'Europa, e che è stato saccheggiato! Concludendo, signora Presidente, ricordiamo Mussari, che da presidente dell'ABI veniva a sollecitare l'attenzione del Parlamento: lui ne sapeva più di noi, perché le truffe le ha

*(M5S)*. Signori, ho scoperto in questi giorni, dopo tanti anni, che Babbo Natale esiste e porta 20 miliardi di regalo alle banche.

Piccola differenza: il debito lo potete fare solo voi che state al Governo e non noi. Noi dobbiamo affannarci a dimostrare come copriamo le spese, mentre voi dite: «Le copro con nuovo debito». Semplice e banale (che stupidi noi che non ci abbiamo pensato).

Rimaniamo su questi benedetti 20 miliardi di euro. Ho i brividi quando sento dire che questi 20 miliardi potrebbero essere spesi per ripatrimonializzare le banche e per interventi molto generici e comunque dopo che c'è stata la suddivisione dei carichi (il cosiddetto *burden sharing*). Questo significa che gli obbligazionisti subordinati sono fregati. restano fregati perché hanno accettato la conversione carta contro carta, cioè obbligazioni contro azioni (quindi i loro soldi li hanno visti la prima volta, quando li hanno dati alla banca, e poi mai più perché adesso stanno solo vedendo carta),

di intervenire con un investimento soltanto da guardone in questo modo? Nessuno. Avete citato il sistema bancario svedese e il caso americano, ma a sproposito perché in Svezia, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito l'intervento è stato così modulato: io nazionalizzo, me la prendo io; guardo cosa c'è dentro, metto in galera quelli che hanno sbagliato e dopo, quando la banca forse l'ho risanata, la vendo. Così ha fatto il Tesoro americano con l'American international group: ha messo 182 miliardi (non si sono infatti posti un limite) e ne è uscito con 22,4 miliardi di plusvalenza. Così ha fatto nel Regno Unito anche la Banca d'Inghilterra con la Royal Bank of Scotland: ha messo

significa aprire i cordoni della borsa del cittadino italiano e metterci dentro non solo le mani, ma tutto quanto il braccio. Basta dirlo chiaramente, però non si può continuare a cercare di toccare l'acqua con un dito, ben sapendo che ci si deve bagnare completamente. un'altra cosa a proposito di questi 20 miliardi di euro. Voi continuate a non citare il convitato di pietra che si chiama Monte dei Paschi di Siena. qui le relazioni trimestrali (terzo e quarto trimestre 2015 e terzo e quarto trimestre 2016). Il problema di tutto sta nel Monte dei Paschi di Siena. Voi state lasciando guardare, state lasciando che l'obbligazionista subordinato ci perda, state lasciando che gli azionisti annaspino e poi, quando tutto quanto sarà finito, deciderete cosa metterci dentro. Ma cosa intendete fare? Almeno su questo qualcosa lo vorrei sentire. Volete andare sul mercato delle opzioni, rastrellare le opzioni e poi prendere tutto l'inoptato, cioè una piccola partecipazione azionaria e non si sa bene come va a finire? Volete entrare più pesantemente? Cosa significa significa ripatrimonializzare? Vuol dire che volete fare un altro aumento di capitale che sottoscrivete integralmente? Queste cose le dovete dire se chiedete 20 miliardi anche perché, come più volte è stato ricordato, voi negate 17 miliardi per il reddito di cittadinanza e poi ne chiedete 20 per buttarli nel calderone del sistema bancario? Non funziona così. Secondo noi questo serve solamente per una cosa, cioè per chiudere il vaso di Pandora aspettando che si apra in un altro momento per permettere al signor Renzi - che è sempre lì, nascosto dietro quella poltrona - di continuare a dire che non è colpa sua, lasciando la patata

proprio sul Monte che ha comprato una banca che valeva 3 miliardi come l'Antonveneta, pagandola 10 - è tutto agli atti - e restituendo ad ABN AMRO i 7 miliardi che ancora la banca Antonveneta aveva di debito. Cioè una banca che valeva 3 è stata pagata 17, quando ancora il Monte dei Paschi di Siena lo sappiamo - dal Partito Democratico e neanche una parola su questo. Ma un po' di rispetto per i cittadini e per i senesi poveracci lo vogliamo avere? Neanche questo vogliamo? Noi continueremo ad insistere in tutte le sedi per l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, ma anche per la vostra perché voi avete proposto una Commissione d'inchiesta sulle quattro banche in risoluzione e poi l'avete lasciata lì. Un altro "spottone" elettorale. Gli italiani non vogliono più sentire parlare di "spottoni" elettorali, vogliono vedere in galera la gente che ha sbagliato. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la principale rivoluzione mancata del Governo Renzi è la riforma dei conti pubblici e la loro messa in sicurezza. Il tema che è oggi all'ordine del giorno doveva essere affrontato prima e non all'ultimo momento, come sta accadendo. Abbiamo assistito a molte manovre sui conti dello Stato per creare facile consenso elettorale, in Italia e all'estero, con una miriade di misure estemporanee. Il debito pubblico vale, a ottobre, 2.223 miliardi di euro, con 116 miliardi in più di quando Renzi è andato a Palazzo Chigi (era 2.107 miliardi nel febbraio 2014). Lo ricordo per l'ennesima volta, perché i numeri sono numeri: con il governo Berlusconi c'erano 316 miliardi di debito in meno, il rapporto debito/PIL era al 120 per cento nel 2011, dopo la legge di bilancio si è attestato al 132,8 per cento. Per effetto della nuova emissione di titoli pubblici per 20 miliardi si porterà ben oltre il 134 per cento, complicando enormemente il piano di rientro verso gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita. inoltre, che la spesa complessiva dello Stato, salita per effetto della manovra di bilancio a 861 miliardi nel 2017, si porterà a 881 miliardi in termini di competenza e, in termini di cassa, si attesterà a 899 miliardi: cifra prossima a 900 miliardi, un altro *record* storico del Governo. Oltre a questa relazione, andranno quindi approvate le opportune variazioni ai totali generali della spesa dello Stato, appena approvati con la legge di bilancio, per il triennio 2017-2019. Va detto, inoltre, che la legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio prevede che ci possano essere scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico in caso di eventi ritenuti eccezionali. deve, però, indicare la misura e la durata dello scostamento, si devono stabilire le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento, si deve definire il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, ma soprattutto - e questo a nostro avviso

Noi siamo sicuramente dalla parte dei risparmiatori, ma non possiamo dimenticare alcuni punti dai quali non si può assolutamente prescindere. Noi ci aspettiamo che il Governo riferisca - e questa è la nostra prima richiesta - in modo rigoroso e dettagliato sull'utilizzo delle risorse. Lo abbiamo detto ieri e lo abbiamo ripetuto oggi in Commissione: abbiamo bisogno che il Governo coinvolga effettivamente il Parlamento nell'*iter* dei decreti e che non lo lasci a margine di un'operazione così complicata e importante per il Paese. Abbiamo bisogno che il Governo definisca un puntuale piano di rientro verso gli obiettivi programmatici e, in ultimo, abbiamo assolutamente bisogno che tutti i cittadini sappiano chi ha responsabilità,

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare è sicuramente di natura straordinaria, sia per l'inedita circostanza che inaugura quanto previsto dalla legge n. 243 del 2016 all'articolo 6, come ricordava il relatore, sia per la portata dell'intervento effettuato: «al fine di tutelare il risparmio e preservare la stabilità economico-finanziaria del Paese, il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario e assicurare la protezione del risparmio». Non siamo oggi di fronte al provvedimento vero e proprio, al decreto-legge o agli eventuali decreti-legge che si occuperanno dei due pilastri di intervento annunciati dal ministro Padoan nella sua audizione, cioè la ricapitalizzazione e il sostegno alla liquidità. Oggi semplicemente autorizziamo, con un provvedimento prudenziale, fino a 20 miliardi di euro di disponibilità che consentiranno di poter valutare varie ipotesi, tutte con l'obiettivo di salvaguardare ulteriormente il risparmio. Le dimensioni di questo intervento, inedite e ragguardevoli, fanno chiaramente intendere come, dopo una lunga serie di sistemazioni ed interventi correttivi e di aiuto al mercato del credito italiano, si sia ora nelle condizioni di dover e poter stendere una rete protettiva che sappia intervenire in modo risolutivo nei casi più critici, pretendendo un completo risanamento e un deciso cambio di pagina rispetto alle gestioni precedenti, di cui i piani di rientro saranno i severi riscontri. È quanto mai evidente che la cifra che viene autorizzata abbia un effetto segnaletico, per adoperare le parole utilizzate in Commissione dal ministro Padoan, ovvero sufficientemente grande da costituire una soluzione per le esigenze fin qua presunte e non eccessivamente grande da far pensare a problemi di dimensioni maggiori di quelli di cui si dibatte ormai da molti mesi. Siamo dunque chiamati ad esprimerci su una questione tanto semplice quanto centrale: con questa autorizzazione ci occupiamo dei risparmiatori o - forse è meglio ricordarlo - continuiamo a occuparci dei risparmiatori dopo averlo fatto con innumerevoli interventi fino ad

sono andati ai risparmiatori e a tutela del risparmio. Quando parliamo di risparmio in Italia facciamo riferimento a cifre importanti, che molti Paesi ci invidiano. Secondo i dati della Banca d'Italia, nel 2015 le attività finanziarie delle famiglie italiane ammontano a più di 4.000 miliardi di euro e tra questi i depositi bancari ammontano a 1.099 miliardi di euro,

quote di fondi comuni per 456 miliardi di euro, valore delle azioni e partecipazioni per 957 miliardi

A fronte di questa enorme ricchezza finanziaria dei nostri cittadini, il totale delle passività delle famiglie italiane ammonta a 918 miliardi di euro, generando così un saldo netto di 3.198 miliardi di euro. Tale livello di risparmio delle famiglie italiane costituisce un'evidente ricchezza per tutto il Paese e va tutelato, secondo quanto prescritto dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 47. La Costituzione stabilisce che il risparmio, «in tutte le sue forme», deve costituire necessariamente oggetto di una specifica tutela da parte della Repubblica e, dopo la riforma del Titolo V, individua proprio nel legislatore statale l'organo competente a disciplinare sia la materia della tutela del risparmio sia, più in generale, quella dei mercati finanziari. È per questo che, anche nel pensiero di uno dei più grandi economisti liberali italiani, Luigi Einaudi, si ammette che lo Stato possa e debba intervenire a sostegno delle banche in difficoltà a tutela del risparmio delle famiglie: i costi del salvataggio - diceva Einaudi - non devono riflettersi sulle finanze pubbliche per non generare e giustificare da parte degli amministratori, comportamenti men che prudenti. Einaudi tuttavia ben presente nelle sue analisi il bene pubblico costituito dalla stabilità finanziaria e dalla salvaguardia del risparmio. Ciò gli fece ritenere del tutto naturale, in presenza di pericoli di corsa al ritiro dei depositi (con conseguenti perdite e fallimenti di imprese e banche), che altri istituti di provata solidità potessero impegnarsi per la garanzia dei depositi e del risparmio raccolto dalla banca in difficoltà, assumendone le attività e tentando di realizzare i crediti. In presenza di masse di ricchezza finanziaria delle famiglie italiane così rilevanti, anche secondo la dottrina giuspubblicistica attuale, «nessun ordinamento giuridico può disinteressarsi a una grandezza macroeconomica di tale rilevanza e portata né può affidare la tutela di quest'ultima di quest'ultima ai soli strumenti privatistici azionabili dalle parti in presenza della conclusione di un contratto». È sicuramente lo Stato, quindi, che può e deve farsi attivamente carico della tutela del risparmio dei cittadini. Inteso come accantonamento di ricchezza, il risparmio diventa un vero e proprio bene pubblico che deve essere assicurato e incoraggiato dallo Stato, che deve garantire il valore sociale della tutela del bene «risparmio», anche e soprattutto in fasi di congiuntura economica sfavorevole. Proprio dal testo dell'articolo 47 della Costituzione emerge il collegamento funzionale tra risparmio e credito e, quindi, con l'attività bancaria, cioè lo strumento necessario per garantire che il risparmio non resti fine a se stesso ma venga produttivamente impiegato. Tutela delle banche in difficoltà significa tutela del risparmio privato delle famiglie e dei cittadini italiani. La Costituzione richiede, ovviamente, non solo la tutela oggettiva del risparmio, ma anche quella soggettiva del risparmiatore, quale consumatore di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi, attore debole che agisce sul mercato. In tal senso, si comprende il collegamento che viene a determinarsi tra il risparmio e la sua origine popolare di cui al comma 2 dell'articolo 47 della Costituzione, secondo cui, appunto, il risparmio va apprezzato soprattutto a partire dal soggetto che ne è titolare, ossia il risparmiatore, e a partire dalla consapevolezza che questa titolarità ha il più delle volte origine popolare e dunque nel lavoro e nei frutti non consumati di questo lavoro. Detto in altri termini, ha origine in una vicenda dell'esistenza delle persone: il lavoro. Ciò costituisce motivo ulteriore che richiede e determina l'intervento dello Stato a tutela del bene «risparmio». Ebbene, onorevoli colleghi, in modo molto responsabile, durante il dibattito in Commissione e anche questa mattina in Assemblea, è emerso un generalizzato senso di condivisione rispetto a quanto oggi andiamo ad autorizzare. Pur in questa condivisione, si sono ascoltate legittime e utili azioni di critica rivolte al passato. Qualcuno sostiene che si poteva fare prima, anche se nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo.

il risparmio e il sistema finanziario. Qualcun altro ha fatto delle critiche rivolte al futuro: chi chiedendo di collaborare nella stesure dei prossimi eventuali decreti-legge (che mi sembra una critica importante e costruttiva), chi suggerendo vincoli di copertura, chi indicando e suggerendo modalità di intervento. Tutto questo mi sembra molto apprezzabile e segno di vicinanza del Parlamento ai problemi dei risparmiatori. Spiace veramente che in questo clima di responsabilità proprio chi si dichiara tutti i giorni vicino ai risparmiatori abbia voluto sfilarsi, addirittura criticando i futuri provvedimenti, di cui non conosciamo nulla per ovvi motivi di plurali possibilità di intervento, ma già sostenendo che ci vorrebbe ben altro. Siamo arrivati in questi casi al "benaltrismo preventivo", e spiace vederlo sbandierare da tradizioni politiche che vorrebbero vocarsi addirittura al Governo del Paese. Siamo in una fase molto delicata, in cui è facile contrapporre la paura e la rabbia alla fiducia e al buon senso. Qualcuno vuole forse vedere i risparmiatori in ginocchio, per poi offrirgli la piazza? Perché è più facile offrire la piazza a chi sta male e a chi è in ginocchio? Al Paese non serve la paura. Non serve la continua delegittimazione delle sue istituzioni pubbliche e private. Al Paese serve ora il buon senso, la solidarietà e l'unità delle forze politiche e del Parlamento. Mai come in questo caso il buon senso si accorderà col senso comune: il costante lavoro di sostegno e ammodernamento del settore bancario (che, ripeto, non ha fatto e non farà sconti ai banchieri) è volto ad sconti ai banchieri) è volto ad un rafforzamento che serve a tutelare i risparmiatori. Ha rafforzato la fiducia nel nostro sistema. sistema. Non si illuda chi crede di lucrare anche su questo provvedimento, di vedere in ginocchio i risparmiatori per poi indirizzarli verso le piazze, perché la fiducia con i nostri provvedimenti

alla prova dei fatti le cose sono estremamente chiare: in questo modo si dice ai cittadini - prima di tutto ai cittadini - che lo Stato è al loro fianco e che non starà a guardare. Perché di questo si tratta con la scelta di questa mattina. Si tratta di dire se lo Stato, il Parlamento, si schiera a fianco dei cittadini e dei risparmiatori o se sta a guardare ciò che capiterà. Il senso di responsabilità, che nelle difficoltà impone di esaminare le azioni possibili e concrete e le loro conseguenze, oggi ci chiede di battere un colpo e di essere presenti. E noi, il Parlamento, dicendo sì questa mattina, rispondiamo a questa chiamata e diciamo in modo molto chiaro ai cittadini: noi ci siamo.

I testi sono in distribuzione. tre osservazioni puntuali. È importante che, al di là, della critica sui tempi di un provvedimento di questo genere, ci sia stata una

sulla necessità, l'opportunità e la convenienza dell'intervento che viene oggi prospettato. Il secondo punto è che mi sembra importante la finalità di questo intervento. Vorrei almeno ribadire, per coloro che, invece, si sono espressi in direzione contraria, che questo intervento non è rivolto a salvare il sistema bancario italiano: non si tratta di salvare alcun sistema; il sistema bancario italiano è solido e non corre alcun rischio di crisi sistemica. Questo non è semplicemente stato ribadito, e dai numerosi *test* che sono stati fatti in questi ultimi due anni. In realtà questo intervento è rivolto verso alcuni casi specifici, ben individuati di crisi, che possono e debbono essere affrontati, come prevedono le stesse norme europee, con strumenti di mercato o, se necessario, con un intervento pubblico. Credo sia importante ribadire tale finalità. Del resto questo intervento è stato poi riconosciuto come necessario da molti degli intervenuti.

perché è concepita nell'eventualità che il mercato possa non farcela a mettere a disposizione le risorse necessarie. Quindi questo provvedimento vuole mettere a disposizione le risorse perché il Governo le possa usare per finanziare delle misure che prefigurino una sorta di rete di sicurezza, di paracadute pubblico. Certo, per evitare il peggio, come si è detto, ovvero secondo le regole europee per evitare che si arrivi alla risoluzione delle singole banche; in questi casi avremmo infatti dei costi enormi non solo per quanto riguarda utenti utenti e imprese, ma soprattutto per i risparmiatori. Quindi questa funzione di rete precauzionale o di intervento è finalizzata ad evitare un'alternativa che, come mi sembra tutti si siano espressi, sia necessario scongiurare. Per concludere, credo che il superamento dello stato di crisi di alcune aziende (che avviene, va ribadito, con interventi che si collocano all'interno delle norme europee, perché è una necessità assoluta, altrimenti non avremmo quei gradi di libertà

potrebbe giovare non solo al complesso delle attività produttive del Paese, ma agli stessi risparmiatori e finalizzato

Chiedo al Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate alla relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Signor Presidente, mi lasci ringraziare i colleghi che sono intervenuti nel dibattito che, tra l'altro, ha contenuto spunti direi non utili ai fini della decisione di oggi, ma assolutamente utili ad inquadrare la questione e a sostenere l'eventuale successivo confronto e dibattito sugli strumenti che eventualmente verranno adottati dal Governo con l'utilizzo

faccio un po' difficoltà a trattare un argomento così importante e rilevante

è qualcosa di indeterminato e non lo dice l'opposizione, lo dice lo stesso Presidente del Consiglio nella sua relazione relazione all'incertezza sulle modalità, sui tempi e sull'entità finanziaria degli interventi da adottare, l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica e il relativo piano di rientro potranno essere dettagliati con i prossimi documenti di programmazione, tenuto conto delle misure che potranno essere effettivamente intraprese». Cioè qui, sostanzialmente, ci chiedete un atto di fiducia e ci chiedete, ancora di più, di dimenticare questi due anni e mezzo, come se in questi due anni e mezzo non fosse successo niente e come se in questo lasso di tempo l'opposizione seria e responsabile di questo Parlamento non avesse già fatto tutta una serie di appunti su come si poteva meglio utilizzare il bilancio dello Stato. Mi viene alla mente l'autorevole intervento del senatore Monti, non più tardi di una settimana fa, quando riprendeva il Presidente del Consiglio su tutti gli atti temerari rispetto all'utilizzo della finanza del Paese, ma questa opposizione aveva detto no alle e questa opposizione non dimentica le frasi del Presidente del Consiglio, quando diceva che fare investimenti sul Monte dei Paschi era un affare. E poi tutta la strategia a coronamento, tutto quello che riguardava il bilancio dello Stato andava affrontato fuori dal contesto della

da una parte alla quale idealmente non appartiene, non possiamo non essere d'accordo sul richiamo

di alcuni ideali liberali soltanto quando si deve fare, ancora una volta, uno *spot*. Noi la tutela dei risparmiatori ce l'abbiamo ben impressa ma, proprio perché abbiamo ben impresso come bisogna operare per salvaguardare gli interessi dei risparmiatori italiani, avevamo fatto ed abbiamo fatto in questi due anni e mezzo tutta una serie di appunti ai quali sempre ed inevitabilmente è stato risposto di no. allora una meravigliosa frase di Martin Luther King, se ci fosse stato il Ministro dell'economia oggi avremmo potuto dire che a noi non fa paura l'ignoranza degli incompetenti, a noi fa paura il silenzio dei competenti. Stamattina avremmo detto al Ministro dell'economia, se fosse stato presente, che lui non poteva non sapere cosa stava accadendo nel bilancio dello Stato e non poteva non sapere anche perché gli Uffici parlamentari di Camera e Senato, in questi anni, hanno sempre dato una dimostrazione di come i conti non fossero assolutamente in linea. Noi oggi non vi accorderemo assolutamente il voto su questo provvedimento, sfidandovi però, perché sappiamo perfettamente che questa discussione ritornerà in quest'Aula con il decreto e allora a quella data e in quel momento noi saremo ben presenti qui in Aula per tutelare gli interessi dei risparmiatori, faremo nostre proposte emendative e vedremo se questo Governo ha deciso di cambiare finalmente rotta rispetto

Signor Presidente, innanzitutto dobbiamo mettere in evidenza che è con un certo imbarazzo che ci troviamo ad affrontare questa discussione, a fronte di una scarna relazione di poche pagine (tre facciate), presentata dal Governo su un tema che è di grande rilevanza: con un'azione del tutto straordinaria, il Governo chiede di stanziare 20 miliardi a debito, contro le regole che sono state inserite in Costituzione.

si è limitato a fare un riassunto di queste tre paginette e non ha detto nulla di più rispetto alla strategia e all'intenzione del Governo. Ancora più imbarazzante è che, al primo atto importante di questo Governo (di questo Renzi-*bis* o Gentiloni, comunque lo si voglia chiamare), si debba affrontare la discussione in un'Aula deserta, soprattutto nei banchi del Partito Democratico che dovrebbe essere qui a difendere questo provvedimento, a fronte di uno stanziamento a debito di 20 miliardi.

"affossa risparmiatori". Si parlava di buona scuola, della riforma costituzionale più bella del mondo. Dietro le parole, voi avete sempre nascosto delle fregature e anche questo provvedimento rappresenta una fregatura. Avete affermato che si tratta di un intervento precauzionale: vedremo se sarà necessario attuarlo. Ma perché tutta questa ipocrisia? Ormai è evidente a tutti che è fallito il tentativo di aumento di capitale di MPS con risorse private ed è evidente a tutti che si concretizzerà questa necessità. L'utilizzo dei 20 miliardi avrà un considerevole impatto sul debito pubblico, soprattutto sul bilancio del 2017. E dopo gli oltre 100 miliardi di aumento del debito nei mille giorni del Governo Renzi, ora il Governo Gentiloni-Renzi prosegue con una richiesta di indebitamento di 20 miliardi, dopo una sola settimana dal suo insediamento. Credo che questo non sia il modo migliore per iniziare. Si tratta solo dell'ultimo di una serie di provvedimenti del tutto fallimentari sia per tutelare il sistema bancario, sia soprattutto per tutelare i risparmi degli italiani. Vorremmo ricordarli brevemente. Ricordiamo la riforma delle banche popolari, impugnata dal Consiglio di Stato, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla sua legittimità; la riforma del credito cooperativo, che è ancora in alto mare; il *bail in* approvato con leggerezza, salvo poi accorgersi delle gravi conseguenze, ratificato come sempre supinamente e poi criticato con un certo timore e un certo imbarazzo, come sempre ha fatto il Governo Renzi. Altro che altro battere i pugni! Avete accettato supinamente dall'Europa parametri insostenibili per il sistema bancario italiano, sbandierando con orgoglio che il nostro sistema era il più solido di tutti e stiamo vedendo in questi mesi e in questi anni quanto solido fosse. fosse. Ricordiamoci poi di quanto poco contiamo a livello europeo: siamo ancora in attesa dell'autorizzazione per utilizzare questo debito di 20 miliardi a fronte di una Germania che anni fa ha investito 260 miliardi per salvare le proprie banche. il Governo italiano attende con trepidazione il via libera non da Bruxelles, ma da Berlino: questa è la cruda verità di questa Europa che voi avete costruito. Bella Europa, complimenti! Avete utilizzato 60 miliardi di denari pubblici per salvare le banche tedesche e francesi che erano esposte con la Grecia e ora dovete elemosinare a Bruxelles e a Berlino l'autorizzazione per stanziare 20 miliardi di euro per le banche italiane: una vera vergogna! Ci sono poi i fallimenti e le responsabilità verso i risparmiatori, che forse sono ancora più gravi. Il decreto salva banche di un anno fa ha messo in ginocchio molte famiglie e risparmiatori: rimborsi lenti, parziali e segnati da continue proteste perché non siete nemmeno riusciti a tutelare tutti i risparmiatori, ma solo una parte.

è stato attuato con un sistema subdolo, per cui, a fronte di investimenti bancari, alcuni istituti bancari si sono rivalsi sui correntisti con prelievi *una tantum* o con l'aumento delle commissioni. Ora voi proseguite questi vostri successi con l'operazione su Monte dei Paschi, che rischia di prevedere altri provvedimenti gravissimi nei confronti dei risparmiatori italiani: l'azzeramento dei risparmi degli azionisti, la conversione forzata dei *bond* subordinati, che riguarderanno 40.000 risparmiatori, e l'aumento del debito pubblico per 20 miliardi di euro senza alcuna garanzia che questa operazione porterà al salvataggio del Monte dei Paschi C'è sicuramente incapacità, ma ci sono anche gravi responsabilità dei vostri Governi di questi ultimi cinque anni. In particolare, le responsabilità sono legate al fatto che più di un anno fa un rappresentante autorevole del Partito Democratico, il senatore Marcucci, annunciò che, a fronte di quel famoso decreto salva banche, sarebbe stata istituita immediatamente una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario: è un anno

volutamente un *iter* farraginoso, lento e fatto di mille audizioni inutili per impedire il varo di questa Commissione. Nell'immediato dell'emozione di quel decreto-legge e del danno che veniva arrecato ai risparmiatori, si annunciò l'istituzione della Commissione e poi si è approfittato del fatto che il tempo che passava, che l'attenzione dei *media* calava e si è fatta la cosa peggiore: insabbiare una Commissione d'inchiesta che era assolutamente necessaria. Siamo stanchi della melina portata avanti dal Partito Democratico, con interventi assolutamente inaccettabili di esponenti del precedente Governo, come il vice ministro Zanetti, che è riuscito ad affermare che la Commissione d'inchiesta doveva essere varata immediatamente e che c'era una irresponsabilità delle opposizioni che non ne acceleravano l'*iter.* La follia allo stato puro: un Governo che aveva la possibilità di indicare alla propria maggioranza una procedura d'urgenza per varare questa Commissione arriva ad accusare le opposizioni di lentezza! La Commissione d'inchiesta avrebbe già dovuto terminare i propri lavori e invece non li ha neppure iniziati, perché nemmeno è stata varata. E mentre i cittadini pagano e i risparmiatori soffrono, abbandonati nella totale indifferenza alla loro disperazione, i responsabili di quelle vicende sono ancora a piede libero, non stanno rispondendo in alcun modo dei propri comportamenti e ricevono compensi e buonuscite milionarie. Ci chiediamo, dopo un anno, cosa avete da nascondere. Cosa avete da nascondere? Perché il Partito Democratico impedisce il varo di questa Commissione d'inchiesta? Ci sono responsabilità politiche da nascondere? Sappiamo che c'è un'interferenza del mondo politico in quello bancario e nel caso del Monte dei Paschi è enorme: nel sistema delle nomine il ruolo del PD è stato sempre decisivo, è evidente a tutti, lo sanno anche gli sprovveduti.

è una delega in bianco. Ma per fare cosa? Non ci è dato saperlo, non lo avete spiegato. Quali garanzie chiederete alla banca per tutelare gli azionisti, gli obbligazionisti, i correntisti, a fronte di questi 20 miliardi? Quali banche se ne avvarranno? Come verranno utilizzati i 20 miliardi? Perché 20? È solo l'inizio? Qual è la vostra strategia, ammesso che ne abbiate una? Non ce lo avete spiegato. Eravamo ben disposti di fronte questa relazione, sentivamo la responsabilità di promuovere questo percorso che era assolutamente necessario per le vostre incapacità di questi ultimi cinque anni. Ma è ormai evidente che voi navigate a vista, pericolosamente e irresponsabilmente. Noi non possiamo e non vogliamo diventare vostri complici in questa triste vicenda. Valuteremo i testi dei prossimi decreti-legge, ma oggi non possiamo votare a favore di una relazione vuota di contenuti. Non possiamo fare un atto di fede: questo Governo non lo merita. La Lega Nord vota contro la relazione del Governo Renzi-Gentiloni. voterò a favore. Non lo faccio da molti anni, ma qui oggi lo farò per evitare la bancarotta della più antica banca del mondo. Ma aggiungo un voto per salvarla anche dall'azione di un Governo che oltre misura è stato cinico e continua ad essere maldestro. Google non perdona e in effetti è così: Adnkronos, 3 ottobre 2016, ore 20,58: Padoan: "Nessuna urgenza su banche". Operazione MPS sarà un successo»; Tgcom24, qualche giorno dopo: «MPS, Padoan: "Nessuna ipotesi di supporto pubblico"».

La domanda che faccio, signor Ministro, è se si tratta di casi ripetuti e seriali di omonimia oppure se è lo stesso Padoan che adesso ci chiede il voto sul testo che discutiamo. È un testo, basta leggerlo, che sembra scritto da Topolino. Dice meno di quello che scrivono i giornali e comunque non dice l'essenziale. Dice che servono almeno 20 miliardi, ma non c'è la correttezza morale e politica di dirci che cosa è successo nel frattempo. Vedete, io credo che la situazione sia ancora più grave di quello che sembra, anche in termini formali. Ma non sono punti giuridici, sono punti potenzialmente tragici, dato il prevedibile sviluppo dei conflitti di giurisprudenza e di competenza che ci saranno. Vedete, l'articolo 81, secondo comma, della Costituzione dispone: «Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico (...) al verificarsi di eventi eccezionali». Le parole chiave sono: "solo", "ciclo economico", "verificarsi legge n. 243 del 2012, citato in epigrafe sul testo che ci avete presentato, ha un contenuto più ampio e probabilmente non conforme al disposto costituzionale. Leggiamolo: si parla di grave recessione economica e di eventi straordinari fuori dal controllo dello Stato. Sulla grave recessione economica credo che sia piuttosto pittoresco il fatto che fino a qualche giorno fa ci raccontavate che eravamo con il segno positivo. Ma il punto più importante - ripeto: costituzionalmente più importante - è quello che riguarda gli eventi straordinari fuori dal controllo dello Stato. Ma vi rendete conto di cosa ci state dicendo? Da una parte dite che il sistema è fondamentalmente sano e dall'altra parte ci dite che c'è una parte fuori dal controllo dello Stato. Questo è allucinante. È sotto il controllo o fuori dal controllo? Siamo in presenza di uno squilibrio sistemico o è una parte del sistema che manifesta criticità? Questo non ce lo dite. E poi, è uno squilibrio già in atto o solo in potenza? Questo è un punto non marginale, ma fondamentale. Tra l'altro, nella relazione richiesta non c'è altro, se non in termini assolutamente generici: non c'è indicazione della misura, della durata, della finalità, dei piani di rientro, degli obiettivi e degli interventi.

tra l'indebitamento e il debito. Mi permetto di far notare che è la somma che fa il totale ed è il totale che alla fine fa il *rating*, dimostrando l'incapacità del sistema per gestire fatti relativamente ordinari, pure essendo importante la salvezza della banca.

(e più o meno ci siamo) e comunque è una fiducia che va chiesta non solo in questa Assemblea, ma nel Paese, a fronte di una realtà sovrastata da una cifra crescente di fenomeni drammatici. In quella sede,

necessaria lucidità e della necessaria capacità nel gestire tutto questo. C'erano già stati gli *stress test*

Ebbene, in quella sede abbiamo detto che, data la natura drammatica dei problemi, era forse il caso, ferme le posizioni politiche, di avviare una discussione comune, nell'interesse nazionale, considerando che la questione in ballo riguarda le famiglie e il risparmio. Non si chiedeva di superare la formazione e la maggioranza di Governo, ma - lo ripeto - si chiedeva di tener conto delle indicazioni che sarebbero venute

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 rappresenta un atto dovuto, ma anche una sorta di cambiale in bianco. Lo stanziamento previsto, fino a 20 miliardi di euro, rappresenta infatti solo una previsione di massima: le cifre effettive dell'aumento del debito conseguente all'emissione di maggiori titoli, a seguito del maggiore indebitamento finanziario, dipenderanno dai successivi provvedimenti che il Governo dovrà assumere, a seconda dell'evolversi di una situazione che non appare predeterminabile *a priori*. Molto dipenderà, infatti, se il piano del Monte dei Paschi di Siena, rivolto al mercato, avrà successo e se vi saranno investitori, sia esteri che italiani, disposti a rischiare le loro risorse per ricapitalizzare una banca da troppi anni trascinata nelle vicende politiche italiane e nei rispettivi giochi di potere. Noi siamo pessimisti, però, perché in questo momento gli investitori hanno bisogno di vedere un Governo forte, stabile e capace

casuali ma strutturali, soprattutto in un momento in cui le opposizioni appaiono molto divise. Abbiamo appena sentito gli interventi della Lega Nord, che si differenziano da quelli di Forza Italia, e questi ultimi si differenziano, a loro volta, da quelli dei 5 Stelle: il popolo del no è frammentato.

(dal Partito Comunista al PDS ai DS) a Siena, sempre e solo governata da una forza politica; alla Banca del Salento, poi Banca 121, che è stata la prima in Italia ad

di Siena, nel periodo in cui presiedeva il Consiglio dei ministri l'onorevole D'Alema. Questi episodi risalgono a un tempo anche anteriore al famoso atto di indirizzo, fatto insolito nel rapporto tra l'ente vigilante e le fondazioni bancarie, emesso dall'allora ministro del tesoro Vincenzo Visco, che aprì la strada alla presidenza di Giuseppe Mussari, uno dei principali responsabili del successivo disastro finanziario. Si sottolineano, invece, i fallimenti degli *stress test* condotti dalla BCE, secondo le regole della nuova vigilanza europea. vigilanza europea. MPS è l'unica banca italiana che ha avuto un riscontro negativo, per cui si rende necessario un aumento di capitale che consolidi il suo patrimonio, tenendo conto, tra l'altro, del volume particolarmente elevato delle sue sofferenze (tra crediti inesigibili concessi agli amici, o meglio ai compagni, agli amici degli amici, incagli e via dicendo) che, che, con un linguaggio più moderno, sono ora chiamati *non performing loans*, che significa fallimento. Si tratta di un inglesismo di cui avremmo fatto volentieri a meno, soprattutto perché questo è l'unico risultato tangibile della tanto decantata unione decantata unione bancaria che, come è noto, avrebbe dovuto comportare ben altri investimenti, come quelli relativi all'assicurazione dei depositi: una garanzia per i risparmiatori. Interventi al momento archiviati, grazie al prevalere delle pregiudiziali dei nostri amici Ma fino a che punto sono amici? Una bella gara, poi, con gli amici francesi, di cui dirò dopo. Naturalmente, un intervento pari a 20 miliardi non riguarda solo la banca senese. Vi sono altri istituti di credito in sofferenza: le due banche venete, le quattro banche locali (Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara), quindi le traversie delle Popolari di Bari. Un quadro, come si vede, complesso e preoccupante, per le eventuali conseguenze di carattere sistemico che la loro crisi potrebbe determinare. Mentre, sullo sfondo, non può essere dimenticato quanto sta avvenendo nei rami alti del capitalismo italiano (e non mi riferisco solo alle vicende che contrappongono Vivendi a Mediaset). Unicredit, la seconda banca italiana, deve ricapitalizzarsi per circa 13 miliardi, e sono in molti a ritenere che questa richiesta segnerà il suo passaggio nelle mani dei francesi i quali, stando almeno ai *rumor* del mercato, punterebbero ancora più in alto: alla conquista di Mediobanca e quindi delle Generali, la signora del capitalismo italiano (mi viene in mente una canzone di Loredana Bertè: «Non sono una signora»). Vedremo nei prossimi giorni se queste sono solo ipotesi e indiscrezioni o se invece rappresentano la manifestazione concreta di quelle scorrerie,

Occorre pertanto, fin d'ora, dare una risposta forte da parte italiana, con un Governo forte, e dimostrare che non si resta impassibili di fronte a propositi di conquista, specie se, come avvenuto nel come avvenuto nel caso di Vivendi, le relative strategie non sembrano essere rispettose delle regole di mercato. Si tratta non di essere a favore o contro un puro liberismo, ma di evitare che l'Italia si trasformi in un'immensa Disneyland, ripetendo gli errori che negli anni passati portarono alla scomparsa delle grandi realtà industriali allora in mano pubblica. Come si vede, la situazione è tutt'altro che tranquilla. Al contrario, i rischi sono rilevanti ed è quindi necessario reagire. Per questi motivi, il nostro voto sulle voto sulle proposte avanzate dal Governo sarà conseguente. Al di là della politica, contano gli interessi nazionali

Noi diamo una fiducia condizionata a questo Governo, diamo un sì condizionato e un giudizio, per così dire, sospeso, pronto a essere rivisto quando le linee di credito saranno state realmente attivate a favore delle singole operazioni. Sarà allora che la valutazione diverrà puntuale e il suo esito tutt'altro che scontato.

la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che il Governo richiede con il voto delle Camere è motivata sicuramente da urgenti profili di responsabilità e straordinarietà. L'adozione di provvedimenti a tutela del sistema bancario e a garanzia del risparmio è motivata dall'evidenza di criticità del sistema creditizio che richiedono misure di sistema in grado di assicurare adeguati livelli di liquidità, il ripristino della capacità di finanziamento e la definizione delle necessarie misure di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sostenute da misure di ricapitalizzazione. Sono questi i punti salienti indicati nella relazione Il principio fondamentale, conforme a tali obiettivi e modalità di intervento, è che sia prevista e riconosciuta la possibilità di concedere la garanzia dello Stato in ordine alle passività degli istituti di credito italiani. Si tratta di un passaggio che corrisponde alle esigenze di decisioni politiche da parte del Governo nei confronti dell'Unione europea dei mercati finanziari e che, a nostro parere, è indispensabile ai fini di una piena tutela dei risparmiatori. Anzi, con il senno di poi, anche rispetto ad altre situazioni che si sono realizzate in passato provvedimenti come questo si sarebbero forse potuti mettere in campo. Si realizza così un'assunzione di responsabilità cui hanno fatto appello le diverse forze politiche, non soltanto di maggioranza. Ci attendiamo, pertanto, un voto che sia conseguente, giacché la misura si configura non come la richiesta di

fino a un importo complessivo massimo di 20 miliardi di euro per il 2017, com'è stato detto, da reperire attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, ha l'obiettivo di affrontare il punto cruciale di crisi del nostro sistema che è, come ormai evidente, l'entità dei crediti deteriorati e la loro strutturale incidenza nei bilanci degli istituti di credito. Non vi è dubbio che vi siano responsabilità di gestione delle banche che non intendiamo né eludere né minimizzare. Ne hanno pagato il prezzo in primo luogo i risparmiatori italiani, la cui platea va ben al di là degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati. È indispensabile, tuttavia ed a maggior ragione, una consapevole valutazione della dimensione ormai abnorme assunta dai prestiti in sofferenza, che dai 199 miliardi al lordo sono attualmente svalutati a 85 miliardi netti nei bilanci dei nostri istituti. Siamo di fronte ad una condizione di sofferenza strutturale, che sarebbe ancor più aggravata da una ulteriore svalutazione dei crediti in sofferenza. Vogliamo affrontare il problema definendo questi interventi come equivalenti ad un paracadute di Stato? Non è così. E così non è stato inteso, non a caso, dall'Unione europea in sede di negoziato. Così non è nemmeno concepito dalla Banca centrale europea, se osserviamo con oggettività i requisiti di capitale richiesti. Gli effetti, o potremmo dire gli obiettivi positivi connessi al sostegno pubblico e che giustificano questa nota di variazione e di ulteriore indebitamento, sono diversi e si intrecciano fra loro: loro: sostenere la ricerca di risorse private i cui esiti dipendono dalla risposta dei mercati e, in alternativa, intervenire salvaguardando la sicurezza; liberare, almeno in parte, le banche sane dagli oneri di mutualità imposti dagli istituti in crisi; evitare la formazione di ulteriori perdite, che determinerebbero una maggiore e sistemica sottrazione di risorse, ancor più ingente, per gli aumenti di capitale che sarebbero comunque indispensabili. Non possiamo oggi sostituirci ai mercati, ad esempio nella risposta che dovranno dare all'intervento privato richiesto da alcune banche a copertura dell'aumento di capitale, ma possiamo e dobbiamo adottare le decisioni politiche e di governo che, se assenti, aprirebbero la via ad una insostenibile crisi di sistema. Nelle crisi di sistema pagano sempre i più deboli: i risparmiatori, le imprese, che vedono e ancor più vedrebbero precluse le opportunità, già ridotte e complesse, di accesso al credito,

titoli di debito pubblico fino a 20 miliardi, in realtà chiede al Parlamento (e di fatto agli italiani) 20 miliardi per il salvataggio del sistema bancario. Qualcuno ha parlato di una cambiale in bianco e potremmo quasi definirla come una richiesta di sottoscrizione di un'obbligazione subordinata.

quali siano le necessarie misure da mettere in campo per la salvaguardia dei risparmiatori. Vi è un'estrema vaghezza o addirittura l'assenza di indicazioni relative alle misure che si intendono intraprendere e quindi è evidente a tutti che questa operazione si sta configurando come un mero e semplice salvataggio,

alla mala gestione degli organi di amministrazione, alla carente attività di vigilanza, che rappresenta un altro elemento. Per questo motivo,

in bianco, al buio, debba attivare gli strumenti in suo possesso, come quello della Commissione d'inchiesta, per indagare, comprendere fino in fondo e accertare le responsabilità della situazione attuale. Per di più noi vogliamo dire con molta chiarezza che adesso si chiede l'autorizzazione per 20 miliardi per il salvataggio delle banche, ma queste somme non c'erano per il terremoto, per il lavoro, per gli interventi urgenti per la povertà. noi avevamo chiesto, anche in modo molto articolato e chiaro, presentando un piano durante la discussione della legge di bilancio (per la verità lo avevamo fatto anche lo scorso anno), di stanziare un punto di PIL, anche a *deficit*, pari a 17 miliardi per far partire un piano

Tra l'altro, recentemente e anche al nuovo Governo, come Sinistra Italiana, avevamo chiesto un intervento pubblico che ritenevamo necessario molto tempo fa;

avremmo mitigato la fuga di correntisti e depositanti. Non lo si è voluto fare quando era necessario e lo si dovrà fare

da conseguirsi attraverso l'acquisizione da parte dello Stato delle obbligazioni subordinate detenute da soggetti non finanziari, che può appunto realizzarsi al prezzo di acquisto e scontando le cedole

con la messa in atto di azioni di responsabilità nei confronti dei vertici passati. Torno inoltre a ripetere che è sempre più urgente l'attivazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta specifica su MPS e, più in generale, sulla situazione del sistema bancario. Oggi infatti sappiamo perfettamente, anche se in quest'Aula non se ne parla,

internazionale potessero arrecare ulteriori danni alla banca e soprattutto ai risparmiatori. Una serie di indicazioni che avevamo dato, chiedendo anche un intervento immediato qualche tempo fa, non sono state poste in essere e oggi ci si

alcuna chiarezza nella relazione sulle linee di intervento che si vogliono adottare. Per noi, la questione fondamentale è la tutela dei risparmiatori e dei posti di lavoro. Pensiamo sia assolutamente necessario intervenire in un altro modo.

in assoluta urgenza perché poi si deve correre a casa a scartare i pacchi di Natale, mentre oggi l'unico pacco che troviamo in Assemblea è la richiesta di delega in bianco. Se siamo arrivati qui è grazie ai mille giorni del Governo Renzi, che sono stati clamorosamente fallimentari per quanto riguarda la gestione del Monte Paschi di Siena

e di parte del sistema creditizio azzerando il *management* responsabile dei disastri degli ultimi anni e separando le banche di affari da quelle di credito ordinario.

per salvare il mondo. Sfido chiunque di voi a prestare a un amico scapestrato un milione di euro per salvare il mondo senza sapere come

al *question time* alla Camera dei deputati, Padoan ha affermato che non si prospettavano per MPS misure di supporto pubblico. E a Sky TG24 il 25 novembre ha rassicurato gli italiani che l'esito del *referendum* non avrebbe condizionato direttamente l'operazione di rilancio della società. Non è vero. Lo diceva cinicamente. Infatti noi sappiamo che, siccome il 4 dicembre il popolo italiano è andato alle urne in massa e ha votato no, i vostri amici della JP

E ancora qui la responsabilità è vostra. La responsabilità è di un Governo che ha tenuto in ostaggio il Parlamento che non ha voluto fare la variazione della Nota di aggiornamento, ha fatto passare al Senato una legge di stabilità con la con la fiducia e, anche lì, ha tolto la possibilità di intervenire. E oggi ci propinate la richiesta di autorizzarvi a spendere di nuovo fino a 20 miliardi senza sapere come. Vergognatevi! Per tutte queste ragioni, per le ragioni di merito che sono state ampiamente e chiaramente spiegate dai miei colleghi e perché, soprattutto, questo Governo continua a non avere una visione ma continua a mettere toppe in modo maldestro sulle spalle dei cittadini, il Movimento 5 Stelle voterà

questo provvedimento ha una prima caratteristica: arriva tardi. E un qualche significato sicuramente c'è perché, naturalmente, nel periodo in cui non è stato emanato la situazione del mercato finanziario e, in particolare, delle banche in Italia ha subìto un ulteriore deterioramento. deterioramento. Nonostante questa situazione, noi ci atterremo a un senso di responsabilità molto forte ed eviteremo ogni polemica, che pur sarebbe assolutamente giustificata da parte di una forza come la nostra. Lo facciamo perché è in ballo in questo momento la tutela del risparmio e, quindi, di centinaia di migliaia di italiane e italiani operosi. Ed è in ballo anche la linfa di un sistema di mercato, che è il sistema bancario. Una grande forza, in un momento come questo, accantona le polemiche e utilizza la sua forza per conseguire quegli obiettivi che ho prima detto: la tutela del risparmio, un rasserenamento del sistema linfatico, del sistema del mercato in Italia. Questa è la ragione per cui noi voteremo a favore di questo provvedimento, la cui natura, però, mi pare necessario ricordare. Questo è un provvedimento di finanza pubblica con il quale il Parlamento autorizza il Governo a andare oltre ai tetti finanziari stabiliti con la legge di bilancio. Dunque, non è ancora il provvedimento di tutela del sistema bancario sul quale, come dirò meglio fra un momento, eserciteremo il nostro diritto di sorveglianza, di critica e, eventualmente, anche di apporto. Lo dico perché questo è un provvedimento di finanza pubblica e, pertanto, ad esso conseguono, con la responsabilità che oggi il Parlamento assume e che noi assumiamo con il nostro voto, alcuni impegni precisi del Governo. che attua questo provvedimento deve avere rigorosamente in questo caso le coperture finanziarie che ad esso sono imposte. Voglio ricordare che oggi si sforano obiettivi determinati con una legge e, pertanto, essi solo con un'altra legge devono essere modificati. E per la modifica di quegli obiettivi ci sono le condizioni e i termini che devono essere rispettati. Il primo dei quali - lo dico subito - è il seguente e saremo attenti su di esso:

quali sono i criteri di copertura cui il Governo si deve attenere nei casi in cui presta la garanzia o nei casi in cui, come questo, addirittura aumenta il capitale. Anche nel caso di sola garanzia è prevista una modalità di copertura, indicata esattamente in quella sentenza ed in tutte quelle successive, che deve essere rispettata. Per cui noi vigileremo affinché l'utilizzo di questi soldi sia adeguato e

cita e sul quale noi - ripeto - dobbiamo attentamente vigilare. Sappiamo perfettamente l'aliquota di incertezza che vige su queste cose, ma sappiamo anche come quell'aliquota di incertezza può e dovrà essere prudenzialmente trattata. Questo è un punto fondamentale al quale noi intendiamo dare particolare rilevanza in questo che - ribadisco - è un provvedimento di finanza pubblica prodromico al decreto che valuteremo nel suo concreto svolgersi. Dunque, attenzione alle coperture e al piano di rientro che nella relazione che oggi approviamo è ancora troppo indefinito, ma che noi riteniamo possa essere ben definito in seguito. Deve però esser fatto nelle prossime sedi.

che noi affidiamo e sul quale intendiamo che il Governo corrisponda, perché è un compito della nostra forza. Al nostro grande senso di responsabilità si associa un grande esempio di controllo e di sorveglianza che una forza di opposizione deve esercitare. Un'altra cosa a cui siamo legati è la seguente. Ciò che noi autorizziamo fino ad un massimo di 20 miliardi è una garanzia o, addirittura, l'assunzione di capitale di rischio. Noi chiediamo allora non solo che quell'assunzione sia fatta con tutti i criteri prudenziali di quando il capitale di rischio è pubblico, come in questo caso, ma che essa sia esercitata con il necessario rigore che i soldi pubblici meritano. L'azionista di maggioranza, ove lo Stato faccia questa scelta in conseguenza del decreto di attuazione del provvedimento odierno, potrebbe essere addirittura l'assunzione del ruolo di azionista di maggioranza di una o più banche. In quel caso deve esercitarlo con tutti i suoi poteri e con la particolare prudenza e il particolare rigore che gli vengono dal ruolo pubblico. Per cui attenzione a tutte le malversazioni di qualsiasi tipo, di qualsiasi natura, da chiunque operate che nel ruolo di esercizio di azionista di maggioranza si possano riscontrare: in quel caso netta e severa dovrà essere l'azione dell'azionista di maggioranza. Vi è però di più. Trattandosi dello dello Stato e di denaro pubblico, è necessario che questa esperienza conduca ad un esercizio di poteri che possa dare la riflessione su alcune questioni che non debbono più ripetersi. Per esempio, sarà utile vedere come è possibile che in capo ad alcuni istituti di credito ci sia una quantità di sofferenze che sono diventate così grandi. Ove mai ci fossero state, al di là delle malversazioni che abbiamo detto vanno punite, delle incrinature del sistema da parte degli amministratori delle banche, ma anche degli enti regolatori, sarà necessario che il Governo, in qualità di colui che rischia, che assume una responsabilità, assuma il potere anche di richiedere la modifica di norme in sede europea e nazionale o la Grazie, signor Presidente. entità che difficilmente possono accumularsi senza un processo sul quale un'azionista ben deve vigilare. In questo caso, infatti, può e deve evitare che tali questioni possano ripetersi, perlomeno nei limiti in cui ciò è possibile. Sappiamo bene che c'è anche una componente strutturale, che è stata la crisi che il Paese ha vissuto, e noi non lo sottaciamo, ma non credo che sia stato solo questo e comunque, ove non fosse stato solo questo, questa funzione deve essere rigorosamente esercitata.

Poiché il Parlamento è chiamato a dare questa approvazione, è necessario che ad esso

oggi, nel votare questo provvedimento, è una fiducia condizionata, nel senso che vogliamo che questi adempimenti siano correttamente e rigorosamente osservati dal Governo nei confronti del Parlamento. Lo riteniamo di assoluta importanza e riteniamo che quando un Governo rischia possa e debba assumere - lo ribadisco - non solo in sede nazionale, ma anche dell'Unione europea, una funzione di partecipazione alla modifica di alcune norme che eventualmente abbiano consentito di portare

a quella normativa, di qualsiasi grado essa sia, che impone la vendita di un qualsiasi oggetto, in questo caso di una banca, ad un termine prefissato, perché è ben noto che a quel termine prefissato il prezzo lo fa l'acquirente e mai il venditore e questo danneggia i risparmiatori. Mi sono limitato a questo, ma potremmo

Grazie, signor Presidente. *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della mozione

per sostenere, ove ve ne fosse la necessità, il nostro sistema creditizio. Il nostro Gruppo voterà a favore anche sulla base della discussione che si è avuta in queste ore, prima nella sede, ieri sera, delle Commissioni bilancio congiunte, poi questa mattina, nella Commissione bilancio del Senato, e adesso nell'Aula del Senato, una discussione nella quale, all'inizio con fatica e poi in modo sempre più forte, la sostanza si è fatta strada sulla forma. C'è stata una forma polemica con la quale la discussione ha avuto inizio e poi, a mano a mano che il merito ha preso il sopravvento, ovviamente il consenso ha cominciato ad allargarsi intorno alla proposta del Governo, una proposta basata sul principio di responsabilità. Vorrei dire che i consensi che si sono aggregati attorno alla proposta del Governo riconoscono che è un atto necessario; qualcuno dice tardivo, ma comunque è un atto assolutamente necessario. Lo voglio dire con rispetto ai colleghi che hanno invece mantenuto un atteggiamento critico e che voteranno contro la proposta del Governo,

con argomenti come sempre pacati, seri e solidi, da parte del relatore, il collega Guerrieri Paleotti: un passaggio all'insegna del principio di responsabilità che dovrebbe essere la cifra fondamentale di questa fase Grazie, È proprio la parola responsabilità la prima parola chiave di questa decisione che stiamo assumendo, una responsabilità alla quale

nei confronti del nostro sistema economico e, in particolare, nei confronti del risparmio che è giustamente e solidamente tutelato dall'articolo 47 della nostra Costituzione.

ciò vuol dire che questi 20 miliardi non sono una cambiale in bianco, come è stato detto, con tono secondo me inutilmente polemico, da parte di alcuni colleghi, ma sono una garanzia di ultima istanza che, proprio per il fatto di essere messa in campo, dovrebbe consentire una soluzione più agevole innanzitutto e auspicabilmente con gli strumenti di mercato. Vorrei rivolgermi al senatore Tremonti che prima ha ricordato in modo un po' malizioso (forse eccessivamente malizioso per chi sa che cosa voglia dire ricoprire le responsabilità di quel Ministero così difficile) che il ministro Padoan si è attenuto a una linea prudente rispettando il mercato: questo diceva mesi fa e questa è esattamente la filosofia del passaggio nel quale ci troviamo. È una linea prudente nel rispetto del mercato,

possa produrre quegli interventi nel mercato che rendano possibile una soluzione a costo zero da parte della finanza pubblica; ove invece ci dovesse essere, per questo o quell'istituto, per questo o quel focolaio di crisi del nostro sistema creditizio, un intervento positivo, l'auspicio è che essere operato secondo i criteri del mercato e quindi produrre addirittura una plusvalenza per la finanza pubblica. Questo è l'obiettivo nel quale ci si muove: un obiettivo - vorrei dire ancora al senatore Tremonti - che a me pare pienamente in linea con la nostra Costituzione, non solo con le direttive europee. lo stesso senatore Tremonti ha ricordato giustamente come l'articolo 81 della Costituzione e, a maggior ragione, la legge n. 243 del 2012, debbano essere letti in sistematico rapporto con l'articolo 47 della Costituzione. E quindi, nel momento in cui si determina un focolaio di crisi, è chiaro che il Governo deve poter disporre di tutti gli strumenti per poterlo affrontare, proprio per evitare che la crisi divenga, poi, qualcosa di incontrollabile e, a quel punto, di irreversibile. Noi stiamo mettendo in campo questo strumento; di questo si tratta, nulla di più, in un'operazione di assoluta trasparenza. Ecco allora la terza parola chiave, con la quale concludo: trasparenza. È stato giustamente chiesto da parte di colleghi superando la loro posizione di opposizione, voteranno a favore della proposta del Governo - che il prosieguo di questo lavoro, ove mai dovessero essere messi in atto decreti o interventi normativi positivi da parte del Governo, da presentare all'attenzione del Parlamento, si svolga con un'assoluta trasparenza e, vorrei dire, anche con uno spirito di forte condivisione, di corresponsabilità parlamentare, rivolto a tutte le forze politiche e, in particolare, rivolto al Parlamento in quanto tale. Io penso che il Senato sia pronto a svolgere questo lavoro. Il Governo, per la voce della ministra Finocchiaro, ieri nella riunione delle due Commissioni V e 5ª di Camera e Senato ha già garantito il massimo

il Governo interviene con una misura economica che ha il sapore del ricatto, mi sia concesso il termine di estorsione morale. L'estorsione, in diritto, è un reato commesso da chi, con violenza o minaccia, costringa uno o più soggetti a fare

dalle norme volute principalmente da Bruxelles, dai dirigenti bancari, collusi con la politica, senza scrupoli e senza etica. Oggi il Governo, con l'espediente dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, chiede di intervenire per fronteggiare «eventi straordinari». Ma quali sono questi eventi straordinari? Con quale denaro? Tagliando ancora il *welfare* o aumentando le imposte? Considerata l'impossibilità di essere uno Stato sovrano, il problema non è intervenire in favore del sistema creditizio italiano, ma di farlo con l'aumento del debito pubblico sotteso a una moneta che non controlliamo, non stampiamo e su cui abbiamo perso ogni sovranità politica ed economica. Prima dell'euro sarebbe intervenuta la Banca d'Italia, ricapitalizzando senza l'aumento del debito per lo Stato; purtroppo l'euro ci impedisce questo intervento. Regaliamo 20 miliardi di euro non per sanare - visto che il prossimo anno, sono sicura, saremo punto e a capo - ma per alimentare quello stesso sistema economico-politico che ha depauperato la forza delle nostre banche, tra cui quella dello storico Monte dei Paschi di Siena. In cambio non riceviamo nulla, neanche i nomi dei responsabili che hanno causato tutto tutto questo, i nomi di coloro che hanno distrutto da una parte il passato dei risparmiatori e dall'altra il futuro dei loro figli. Ecco perché voterò contro: a questo punto non posso essere complice di questa estorsione. Esprimo il mio voto contrario per dignità,

Signor Presidente, prendo la parola con un certo imbarazzo, perché a ruoli invertiti anche noi avremmo presentato un provvedimento per salvare i correntisti e i clienti delle banche. tuttavia, accettare che tutto questo avvenga senza una forte critica a chi ha gestito il sistema bancario e, in modo particolare, il Monte dei Paschi di Siena.

Alcuni anni fa è stato in qualche modo crocifisso Mussari. Per carità, meritava tutte le critiche che gli sono state fatte, è intervenuta la magistratura, che farà il suo corso (non mi interessa); ma sono passati diversi anni e da allora il Monte dei Paschi non è riuscito a invertire questa rotta disastrosa. Eppure nel 2015 ci era stato detto che il sistema bancario andava bene e che tutto funzionava bene. Non mi pare. Questo provvedimento è indispensabile, me ne rendo perfettamente conto; ma, così com'è stato presentato, non mi consente di votarlo. E siccome non sono abituato a votare in dissenso o comunque in maniera difforme dal Gruppo al quale mi onoro di appartenere, non parteciperò al voto.

che impatta decisamente sull'interesse della nazione e sulla tutela dei correntisti la quale, peraltro, avrebbe potuto essere anche meglio specificata. Ma esso ha anche un significato politico,

Un giudizio sul pressappochismo di impegni presi dall'ex Presidente del Consiglio, acriticamente assunti dal Ministro dell'economia e comunicati con troppa leggerezza alla pubblica opinione. Un giudizio sul perché alcune soluzioni alternative a quelle che facevano capo al ruolo centrale di JP Morgan non sono state mai prese in considerazione. Un giudizio sul fatto di non aver mai fugato l'impressione - che ora è più di un'impressione - che tutto ciò sia accaduto perché vi sia da coprire un passato che non passa.

Signor Presidente, senza ripetere le motivazioni già esposte dal senatore Matteoli, che condivido fino in fondo, e in gran parte quelle esposte dal senatore Quagliariello, annuncio che non parteciperò al voto.

Ricordo che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pertanto la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo.

Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla cosiddetta

è oggetto di opere di escavazione all'interno del Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV), il cui fine sarebbe ottimizzare la gestione delle acque, ma suscita preoccupazioni nella popolazione per per come viene effettuato, soprattutto nei Comuni dell'alta padovana, come Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Piazzola sul Brenta. Sono questi solo alcuni dei Comuni in cui si sono sviluppati spontaneamente dei comitati, come il comitato "Giù le mani dal Brenta", il "Gruppo ambiente Carmignano" e il comitato "Brentana Guardiana", che hanno fornito un contributo fondamentale. Ci sono delle violazioni in atto. I lavori di scavo sono partiti già il 29 marzo, con tanto di mezzi cingolati, nonostante l'accordo sottoscritto dai Comuni ne proibisse l'uso e la zona dei lavori sia soggetta a vincolo dell'Unione europea, atto a proteggerne la biodiversità, per cui da marzo ad agosto non si potrebbe effettuare lavoro alcuno. Per contro, i progetti di ricarica della falda, da farsi prima dell'effettivo inizio dei lavori, sono stati lasciati a data da destinarsi. presentati tre esposti tra il 2015 e il 2016 ad opera dei comitati, tre richieste di incontro nel 2016, che hanno prodotto solo la promessa di essere ricevuti per la consegna delle firme della petizione, una Il Movimento 5 stelle si è attivato ad ogni livello. In Veneto in data 30 marzo 2015 l'allora consigliere di Cittadella Loris De Poli fu il primo Il testimone oggi è passato a Sabrina Meneghello, consigliere di Piazzola sul Brenta, insieme a Manuel Brusco, consigliere regionale. Il collega deputato Brugnerotto, in data 9 maggio di quest'anno, ha depositato un'interrogazione al ministro Galletti, rimasta ancora senza risposta. L'eurodeputato Marco Affronte ha sollevato la questione presso le sedi di Bruxelles. Voglio dunque riportare qui in Assemblea la voce e le domande dei cittadini. Qual è il vero obiettivo che porta, rispetto ai pozzi di Camazzole, a distruggere un *habitat* naturale per costruire in alveo (zona assolutamente non idonea) cinque nuovi pozzi non necessari? Sui progetti di escavazione a Santa Croce Bigolina, perché mettere a rischio la sicurezza idraulica dell'area estraendo un quantitativo di ghiaia dall'alveo del fiume per volumi superiori al valore delle opere pubbliche che le imprese appaltatrici metteranno in opera? Qual è il vero obiettivo delle opere di compensazione che comportano scavi di centinaia di miliardi di metri cubi di ghiaia? Quali misure si intende adottare per il progetto «Democrito», che ad oggi non è stato finanziato dalla Regione Veneto? Si tratta di 18 milioni di euro non attuarlo significa compromettere la ricarica delle falde acquifere. Infine, quali garanzie abbiamo che le cave da cui si procede con l'escavazione non vengano utilizzate per scopi che minaccino l'ambiente

Presidente, questo Governo riesce a trovare 20 miliardi per salvare le banche private che la politica ha spolpato in questi anni. Vedremo cosa sarà in grado di fare per salvaguardare 400 posti di lavoro e indotto presso le quattro aziende Sanac che operano in Italia. Sanac fa parte del gruppo ILVA:

fa la sua produzione per circa il 60 in quella direzione. ILVA non paga Sanac, Sanac non paga i fornitori e diventa insolvente, pur essendo un'azienda sana. Oggi è commissariata ovviamente, è in amministrazione straordinaria. fare - si procederà a una vendita scorporata di queste aziende satelliti di ILVA, ci troveremo di fronte a una frammentazione, uno spezzatino dove chi acquisterà senza dubbio lo farà nell'ottica del massimo ribasso e con le tutele nei confronti dei lavoratori senz'altro peggiorate. come succede, chi oggi viene a fare *shopping* in Italia si prende la tecnologia *know how*, smantella e, dopo poco tempo, arrivederci. Il giorno 12 dicembre c'è stato un incontro al MISE con i lavoratori, la proprietà, i commissari. Si chiede sicurezza di continuità di forniture a ILVA e salvaguardia

ore di sciopero e un presidio in Regione Toscana. Il Movimento 5 Stelle ha presentato in Regione una mozione approvata all'unanimità in cui si chiede che il Governo si attivi per bloccare la messa in vendita separata entro il 31 gennaio e si possa trovare una soluzione condivisa e rispettosa del diritto alla continuità e alla certezza del lavoro. La crisi che coinvolge la siderurgia è il frutto della mancanza di una visione nazionale sul futuro dell'acciaio in tutta Italia. Chi ci rimette alla fine sono sempre i lavoratori e le loro famiglie. Sappiamo che la vertenza Sanac è sul tavolo della vice ministro Bellanova. Abbiamo depositato un'interrogazione per i lavoratori Sanac. Chiediamo pertanto a questo Governo di prodigarsi celermente per dare risposte rassicuranti e far passare buone buone feste a così tante famiglie preoccupate. Chiediamo ai ministri Calenda e Poletti atti concreti e possibilmente in tempi utili. *(Applausi